Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», il cui elenco dei componenti è stato pubblicato in allegato al Resoconto della seduta di giovedì 18 luglio 2024, è convocata giovedì 1° agosto prossimo, alle ore 8,30,

una nuova finestra"). Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport» (1206).

buon compleanno, gli auguri più affettuosi da parte di questa Presidenza.

per Giorgia Meloni Palazzo Chigi val bene un'abiura, anzi più abiure. È lontano il tempo (correva l'anno 2014) in cui Giorgia Meloni, allora segretaria di un partito di opposizione, attaccava il Presidente del Consiglio in carica, incidentalmente Matteo Renzi, accusandolo di essere amico della Cina e della sua concorrenza sleale. Meno lontano, signora Presidente, il tempo (era il febbraio 2021) in cui l'allora unica *leader* dell'opposizione attaccava "il regime comunista di Pechino per gravi violazioni della libertà di stampa". Ci sarebbe da sorridere amaramente, visto che la Presidente del Consiglio ha scelto proprio la Cina come luogo e quinta teatrale per il suo attacco ai giornali da lei definiti di opposizione. Presidente, nella prima lettera cinese di Giorgia ad Ursula si propone come mediatrice tra Pechino e l'Unione europea, peraltro con un senso delle proporzioni e del proprio peso politico un po' da vertigini, visto che prima Olaf Scholz e poi Emmanuel Macron l'hanno preceduta in terra cinese e Xi Jinping è andato in visita ufficiale in Francia, ma non è venuto in Italia. Ma, al di là di questi aspetti, dalla Cina, proprio da quella Cina delle gravi violazioni della libertà di stampa, il nostro Presidente del Consiglio si è peritato di chiamare per nome le testate a lei sgradite. Ecco, non vorremmo che l'aria di Pechino in materia di pluralismo l'avesse contagiata. poi un tema istituzionale e politico di primaria grandezza, che pongo all'attenzione dell'Aula, chiedendo formalmente un'informativa della Presidente del Consiglio. dove si è discusso in Parlamento della conversione a "U" della *Premier* sulla Cina? Dove e quando è stato dato mandato alla Presidente di firmare un non meglio precisato piano triennale di cooperazione industriale? siamo usciti dalla Via della Seta, cui noi eravamo favorevoli, senza un dibattito parlamentare, alla chetichella, così. Ora ci sono dei *dossier* delicatissimi in ballo, giova ricordarlo. La Cina sostiene la Russia nella drammatica vicenda ucraina. *(Applausi)*. La Cina sostiene l'Iran e i suoi *proxies*, di cui abbiamo avuto nei giorni scorsi, purtroppo, ancora dimostrazione. La Cina tiene in vita il regime comunista della Corea del Nord. La Cina fa esercitazioni militari con la Bielorussia. La Cina, nelle scorse ore, si è appena congratulata con Maduro. Domanda: di questo se n'è parlato a Pechino? La Cina esporta, facendo *dumping*, con tecnologie rubate all'Occidente, usa il lavoro forzato, viola i diritti umani. Domanda: di tutto questo se n'è discusso a Pechino? La Cina è proprietaria di industrie sulle reti di quinta generazione presenti in Italia, che possono pregiudicare la nostra sicurezza. Domanda: se n'è discusso a Pechino? Per non parlare dell'intelligenza artificiale dell'*automotive*, di cui leggiamo sui giornali si sarebbe discusso. Insomma, abbiamo avuto un'immagine di eccessiva remissività e velleitarismo; un'immagine che

lasciando sulla spalla laterale l'incontro con la presidente del Consiglio Meloni. Colleghi, per i cinesi noi siamo laterali rispetto a Timor Est. Ce n'è abbastanza, signora Presidente, affinché la Presidente del Consiglio venga a riferire in quest'Aula.

Al tempo stesso, però, sappiamo benissimo che questa sfida, questo Piano, non appartiene soltanto al Governo e alla maggioranza, ma appartiene a tutti gli organi istituzionali, compreso il Parlamento.

Piano nazionale di ripresa e resilienza. Attraverso il PNRR molte delle difficoltà e delle emergenze del nostro Paese possono e devono essere risolte: quel Piano è nato proprio per questo, ad esempio per affrontare i problemi della siccità.

di indirizzo, vigilanza e controllo per cercare di affrontare e risolvere meglio i problemi per la spesa reale del PNRR. Solo alcuni giorni fa si parlava, per esempio, del fatto che ci sono ritardi eccessivi

è relativa a crediti di imposta sia del superbonus sia della Transizione 4.0 e questo è un problema anche per le anche per le prossime rate del PNRR, perché se non andiamo avanti con la spesa nel 2004 e nel 2025, non avremo l'erogazione delle rate, dovremo un'altra volta rimodulare e riformulare gli obiettivi.

perché quello a cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni è effettivamente singolare. Non è mai accaduto, cioè, che venga indirizzata una lettera da parte del Presidente del Consiglio nei confronti della Commissione europea per commentare un *report* che, come tutti i *report* dello stesso tipo, è indipendente e ha a che fare con un vincolo che la Commissione europea si è data, cioè quello di monitorare l'evoluzione dello Stato di diritto, su quelli che possono essere commenti, tendenze, evoluzioni che possono riguardare la vita democratica. È un tema che ci riguarda tutti, che non individua responsabilità personali, ma che interpretare come un attacco politico evidentemente espone anche il nostro Paese

a un *report* che ha a che fare con l'evoluzione del pluralismo, della libertà di espressione, del rapporto fra poteri e mezzi di comunicazione, fra potere pubblico e servizio pubblico radiotelevisivo, e si risponde

una sorta di reazione mediatica di altre testate contro altri giornalisti, questa forse è la dimostrazione che c'è quantomeno un clima che non è di serenità e di reciproco di reciproco rispetto, che sono esattamente quei principi e quei fondamenti che quando parliamo di Stato di diritto chiamiamo in causa. L'anno scorso qui posi questo tema rispetto alle nomine relative alla RAI e in particolare alle annunciate dimissioni

cercare un sostegno esterno per la difesa della democrazia. Noi vorremmo un sostegno interno da parte del Governo e delle forze di maggioranza, per unirsi nel contrasto alla disinformazione, nella difesa dell'indipendenza, del pluralismo e dell'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo, anche rispetto alla circostanza nella quale qualcuno

vanno discusse e confrontate. Si può anche discutere duramente, come facciamo nelle diverse Commissioni, ma tutto possiamo fare tranne che attribuire ad un documento indipendente che viene dalla Commissione europea il carattere di attacco politico.

di avere il consenso. Una democrazia non si giudica per la qualità e la quantità del consenso che riceve, ma per la capacità - diceva Ronald Dworkin - di tollerare il dissenso. Questa è la democrazia: la capacità di tollerare il dissenso, la capacità di dare spazio al pluralismo e alle voci critiche, senza pensare che questo sia un attacco alla democrazia. Perché quando questo avviene è esattamente il capitolo 1 del libro "Attacchi allo stato di diritto".

11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali" (1162)

il decreto-legge in esame reca in primo luogo una serie di modifiche alla disciplina della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023. Esso contiene poi una disposizione relativa agli uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo a seguito del sisma del 2009 e altre misure in materia di protezione civile, nonché infine disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Nel corso dell'esame il Governo ha presentato un emendamento che ha trasfuso, all'interno del suddetto decreto-legge, il contenuto del decreto-legge n. 91 del 2024 recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e coesione. I primi sei articoli riguardano la ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023. L'articolo 1 autorizza il commissario straordinario a concedere nel limite di spesa di 210 milioni di euro contributi per i danni ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati in seguito agli eventi alluvionali. Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un emendamento che circoscrive l'ambito di applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo agli eventi sismici verificatisi quell'anno, ai contributi per i soli beni mobili registrati. L'articolo 2 prevede la concessione di contributi a cittadini e imprese per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative o di immobili immediatamente disponibili nel caso in cui non sia possibile provvedere alla ricostruzione nello stesso luogo. L'articolo 3 prevede che il commissario per le azioni di controllo possa avvalersi, oltre che della propria struttura di supporto, anche di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettive, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo dei contributi pubblici. L'articolo 4 proroga la durata del mandato del commissario straordinario alla ricostruzione dal 30 giugno al 31 dicembre 2024 e prevede semplificazioni per l'assunzione di personale da adibire ai procedimenti di ricostruzione da parte degli enti locali. L'articolo 5 estende il novero dei soggetti che possono essere individuati quali soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, includendovi le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organismi *in house*, gli enti pubblici economici, le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllate, le aziende sanitarie locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un emendamento che riguarda le nomine dei responsabili unici di progetto da parte dei soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. L'articolo 6, conseguentemente al 5, al fine di intervenire celermente anche sul dissesto di versante nei territori collinari e montani, che spesso insistono su proprietà di piccoli comuni oppure su proprietà private, affida gli interventi di ripristino delle infrastrutture ferroviarie e di contrasto al dissesto di versante incombente sulle stesse e sulle aree contigue al gruppo FS, nel limite massimo di 255 milioni, e gli interventi di ripristino delle infrastrutture stradali e di contrasto al dissesto di versante gravante sulle stesse e sulle aree contigue ad ANAS. L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, interviene sulle modalità di individuazione dei soggetti incaricati delle attività di raccolta e trasporto dei materiali di scarto. L'articolo 7 riguarda il sisma del 2009 e specifica che nelle risorse statali che il CIPESS può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possano rientrare anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione. Nel corso dell'esame in Commissione sono stati inseriti due commi aggiuntivi; il primo riconosce un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento architettonico, mentre il secondo riguarda la destinazione delle risorse per la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata stanziate dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013. L'articolo 8 consente di ricorrere alle risorse di cui all'articolo 1, comma 448, dalla legge di bilancio del 2022, anche per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza nazionale, verificatisi negli anni 2022 e 2023, per i quali non siano stati previsti finanziamenti con norma primaria. L'articolo 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, proroga fino al 17 settembre 2025 lo stato d'emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nelle Marche. L'articolo 9 estende per un ulteriore quinquennio a favore dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo l'efficacia temporale del regime speciale di reclutamento del personale previsto per gli enti pubblici di nuova costituzione. Come ho anticipato prima, nel corso dell'esame in Commissione sono stati inseriti due nuovi capi: il nuovo capo II-*bis* reca ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Queste misure si innestano nell'ambito di un percorso già avviato con il decreto-legge n. 140 del 2023 e si sono rese necessarie in seguito all'ulteriore evento sismico del 20 maggio scorso, per il quale è stato dichiarato lo stato di mobilitazione. L'articolo 9-*bis* disciplina l'attuazione e il finanziamento delle misure relative al patrimonio edilizio, anche privato, localizzato nella zona di intervento, delimitata in data 27 dicembre 2023 e oggetto di un piano straordinario. La zona comprende parte dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, con una popolazione di circa 85.000 persone e un numero stimato di 15.000 edifici. Inoltre, disciplina l'attuazione del finanziamento delle misure relative alle infrastrutture di trasporto e dei servizi essenziali prioritari. L'articolo 9-*ter*, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prevede che sia nominato un commissario straordinario, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2027. Viene conseguentemente abrogata la disposizione della legge n. 219 del 1981, che aveva attribuito al Presidente della Regione Campania il ruolo di commissario straordinario per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, prevedendo che entro sessanta giorni trasmetta trasmetta al Governo una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento e dettando disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dal programma suddetto. L'articolo 9-*quater* reca misure di semplificazione e accelerazione derogatorie per l'attuazione degli interventi. L'articolo 9-*quinquies* prevede che il commissario straordinario esegua interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici danneggiati e sgomberati per inagibilità, nel limite di 15 milioni di euro per il 2024, proprio in seguito all'evento sismico del maggio scorso. Nelle more, la Regione Campania potrà avvalersi dell'accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati a uso scolastico. L'articolo 9-*sexies* autorizza la Regione Campania ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata. Nel corso dell'esame in Commissione, oltre a chiarire che l'abitazione principale dev'essere abituale e continuativa, sono stati aumentati gli importi del Fondo per le emergenze nazionali che possono essere destinati a coprire gli oneri derivanti dall'articolo in esame. L'articolo 9-*septies* prevede che entro novanta giorni la Regione Campania adotti gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico e ad evitare l'incremento del carico urbanistico. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione, sono vietati il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale. L'articolo 9-*octies* disciplina la procedura per l'adozione di un programma di interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto di contributi, una volta conclusa l'analisi di vulnerabilità sismica. L'articolo 9-*nonies* introduce contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica di riparazione del danno sempre in seguito all'evento sismico del 20 maggio scorso, a favore del patrimonio edilizio privato, stanziando a tal fine 20 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Nel corso dell'esame in Commissione è stato chiarito che il contributo di cui all'articolo in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef dei beneficiari. L'articolo 9-*decies* proroga fino al 31 dicembre 2025 la durata della struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo dipartimento della protezione civile. L'articolo 9-*undecies* prevede che il CIPESS assegni alla Regione Campania la somma complessiva di 388.557.000 euro per il completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del L'articolo 9-*duodecies* riguarda gli interventi successivi al sisma del 2016 e dispone la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione e introduce un nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. L'articolo 9-*terdecies* differisce al 2025 la decorrenza delle nuove assunzioni di personale non dirigenziale per tutti gli enti territoriali del Mezzogiorno e del Dipartimento delle politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e rimodula conseguentemente il nuovo quadro finanziario. L'articolo 10 destina risorse straordinarie a Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del vertice G7 L'articolo 11 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, in virtù della quale si deve intendere che le attività svolte dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, detta disposizioni in materia di valutazione delle richieste di contributo a carico dello Stato per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale. Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.

"ricostruzione" al nostro esame penso tocchi nella carne viva del Paese i tanti drammi che abbiamo subito in questi anni e sono azioni che abbiamo visto, ognuno di noi parlamentari, sul territorio in maniera molto forte.

hanno colpito nei sentimenti. Il mese di maggio del 2023 ha portato via quindici persone: 3 da Forlì, 4 dalla provincia di Cesena, 7 dal Ravennate e uno dal Bolognese. Ci sono state decine di migliaia di sfollati, ma questa alluvione non ha portato via la dignità dei romagnoli. Non smetteremo mai in quest'Aula di portare avanti i temi per non far spegnere le luci sull'argomento dell'alluvione che ha colpito il nostro territorio. Queste famiglie arrivano fortemente ai parlamentari e ai sindaci dei propri territori; a noi hanno portato tanti emendamenti, rispetto a tanti temi che in questo anno sono stati dimenticati e che abbiamo portato all'interno di quest'Aula, in particolare all'interno di questo provvedimento. Un'azione politica molto importante è stata fatta proprio da uno dei sindaci del territorio di Ravenna, Michele De Pascale, che ha convocato tutti i parlamentari del territorio portando emendamenti specifici e noi come forze politiche di opposizione abbiamo lavorato insieme per attenzionare il Governo. Il problema che abbiamo visto la maggioranza fare passerelle sulla nostra terra, venendo con gli scarponi, passando con gli elicotteri, venendo con Ministri che hanno detto che il Governo non è un bancomat. state manifestazioni, in cui i cittadini sono venuti in piazza a protestare, sotto il comune di Forlì in particolare, e sono stati transennati, messi alla berlina e addirittura chiamati facinorosi, perché contestavano che a un anno di distanza ancora non si sia visto nulla. C'è stata quella particolare comparsata a Forlì della presidente Giorgia insieme alla von der Leyen: probabilmente questo tipo di passerella insieme non la vedremo più, visto l'epilogo che c'è stato in Europa che ha sancito che non contiamo niente e che siamo isolati per la nostra incapacità politica. qua da Roma si fanno racconti, si promettono cose sul territorio della Romagna e non è stata versata una lacrima, lì si sono rimboccati le maniche per risolvere i problemi da soli.

le persone sono tornate a lavorare senza motori, macchine e biciclette. Hanno trovato il modo di andare a lavorare in egual maniera. Nei Comuni sono sono state riaperte le scuole. Si è ricominciato ad insegnare ai ragazzi senza più le scuole di prima e senza più le classi di prima. Le famiglie hanno continuato a cucinare, hanno continuato a lavorare, senza più le loro cucine e senza più gli spazi domestici che avevano prima. Gli agricoltori, senza più gli strumenti, hanno continuato a produrre sul territorio, in eguale maniera rispetto all'anno precedente. I parroci, con le chiese devastate, hanno continuato a fare le proprie funzioni religiose, come se non fosse successo niente, come se fosse tutto Questa è la Romagna, questo è il sudore dei romagnoli, con lo stesso identico sorriso. Addirittura, abbiamo dimostrato una rabbia composta con la pacifica manifestazione fatta durante il *Tour* *de France*, durante la quale i cittadini alluvionati, arrabbiati, vestiti di giallo, hanno promosso un *tour*

che questo Governo deve comprendere. A questi emendamenti, che ripresenteremo in Aula oggi, riceviamo, però, sempre le stesse identiche risposte.

altro della vostra incapacità. È stata data la colpa ai benzinai, all'Europa, al superbonus, per il problema dei conti del Governo.

perché, con 23 fiumi esondati contemporaneamente, 13 fiumi a livello di allarme, 80.000 frane, 772 strade chiuse, dal 1° al 17 maggio sono state aperte

In Romagna non c'è stato nemmeno il tempo di versare una lacrima, ci si è rimboccati le maniche immediatamente. I mesi passano e la rabbia la rabbia sta crescendo sui territori. Non è sulle prime pagine dei giornali, ma è una rabbia che cresce continuamente. Abbiamo dovuto attendere due mesi un commissario straordinario cui avete dato gli strumenti un mese successivo: questo è inaccettabile! La nomina di un commissario straordinario è inaccettabile. Sul territorio non si fa campagna elettorale. Noi ricordiamo perfettamente quello che è stato detto. Non so se fosse, appunto, un *trip* elettorale, ma avete parlato di ristori al 100 per cento. Io spero che non sia come nei classici video che Giorgia proponeva, dove andava dal benzinaio e tagliava le accise. Abbiamo parlato continuamente della necessità di beni immobili e, finalmente,

che non è quantificabile per quello che è successo. Io le immagini le ho negli occhi, ma penso anche molti colleghi e tanti di voi. Quando un fiume di fango entra dalla porta e esce dalle finestre dell'altra stanza;

Avete trovato fondi per tutto; anzi, non abbiamo trovato come Parlamento fondi per niente,

Concludo ricordando una cosa e ringrazio come sempre la Presidente per il tempo che mi ha concesso. Concludo ricordando a tutti che chi ha messo sul territorio il proprio impegno sono state le Forze dell'ordine, la Protezione civile, l'Esercito, la Croce Rossa, in particolare i volontari e soprattutto i sindaci dei territori. Continuare a considerare i sindaci come colpevoli di non riuscire a realizzare quello che il Governo deve fare è vergognoso. C'è però una storia positiva nella Romagna e tutti la dobbiamo ricordare: sono stati i giovani che sono venuti ad aiutarci nel momento più difficile;

*baby-gang* a manganellarli quando vanno alle manifestazioni, dal pensare di fargli fare la leva obbligatoria al mettere nei consultori le associazioni pro-vita, tutti quelli che protestano per l'ambiente vengono arrestati perché fanno atti estremi. Questa è un'azione che sconvolge l'ordine di questo Paese. I giovani devono essere i primi ad essere tutelati e gli ultimi ad essere criticati. Sono stati loro i primi ad arrivare in Romagna e gli ultimi ad andare via. Sono loro che la Romagna ringrazia, non questo Governo fatto di chiacchiere e distintivo. Signora Presidente, il senatore Croatti ha ricordato i giorni drammatici

Ci si aspetterebbe che, in un intervento urgente sulla post-calamità, quel "*post*" sia riferito all'urgenza del periodo. Qui invece è passato molto tempo. Noi di solito ci lamentiamo di una decretazione d'urgenza inopportuna, impropria, strumentale. In questo che è urgentemente in ritardo, perché sono state fatte delle promesse a cittadini, famiglie e imprese che non sono state rispettate. La proposta che si fa in alcuni casi di avere 6.000 euro per un ristoro rispetto a un dramma familiare, economico, patrimoniale di famiglie e imprese è veramente un elemento ridicolo. Qui non c'è da speculare, non c'è da fare strumentalizzazione politica, perché questi sono eventi questi sono eventi drammatici, che ovviamente non hanno colore politico, né dal punto di vista del momento immediato del soccorso, né dal punto di vista dei rimedi e dei ristori.

Meloni), non ci vanno come rappresentanti di un partito e neanche di una maggioranza di Governo; ci vanno come istituzioni, *(Applausi)* per far sentire a quella popolazione che non sono rimasti soli, che ci sono le istituzioni al loro fianco, esattamente in quei momenti, nei momenti in cui non resta nulla, non resta una casa, non restano le cose che ti hanno accompagnato per tutta la vita, non restano le imprese, non restano le strutture. Lì c'è una solitudine rispetto alla quale rispetto alla quale soltanto un'istituzione può dare l'idea di una vicinanza: non siete soli. Noi oggi però - come ha detto il collega prima - con questo decreto-legge non stiamo dando questo messaggio. Stiamo dicendo piuttosto il contrario: siete soli, perché noi non siamo stati in grado di varare misure significative che effettivamente possano agire da ristoro per quello che è successo. Questo non è un tema di strumentalizzazione politica. Noi potevamo sederci insieme, ci sono state riunioni dell'8a Commissione alle quali abbiamo partecipato, con moltissimi emendamenti discussi; altri vengono ripresentati in Aula, perché sono stati bocciati. Nelle discussioni che abbiamo avuto siamo rimasti molto perplessi, perché molti di questi emendamenti avevano osservazioni sia in termini di spesa e di oneri (ma gli oneri erano stati indicati, si tratta di fare delle scelte politiche, come è stato detto),

uno che mi ha abbastanza impressionato: il rifiuto della digitalizzazione per la trasparenza degli appalti, che è un tema che di per sé dovrebbe interessare tutti, perché aiuta la tracciabilità della spesa di risorse pubbliche. Anche quell'emendamento è stato bocciato. Ma in generale, anche se qui si parla di post-calamità, quello che manca, quello che noi tutti dovremmo fare insieme in questo Parlamento è renderci conto che il mondo è cambiato, che è cambiato il clima, che non siamo più davanti a variazioni e calamità occasionali, ma siamo purtroppo entrati in un contesto drammatico di ripetizione, rispetto al quale occorre una legislazione profondamente diversa: la creazione di un fondo di sostegno per le calamità, qualcosa che possa essere rinnovato costantemente e che sia immediatamente disponibile, proprio per attivare misure immediate quando si verificano calamità. Questo non è avvenuto. C'era l'occasione di farlo in questo contesto, anche con le risorse esistenti, con l'idea poi di fare un fondo che potesse essere rifinanziato nel corso del tempo. Questa visione, questa capacità di unire il Paese in un interesse comune, per stare vicino alle popolazioni, questo decreto non le persegue. Ci sono altre questioni che emergono. È stato citato il caso dell'Emilia-Romagna (ne parlerà più diffusamente il collega Manca). Ma anche l'intervento sui Campi Flegrei (di cui parlerà la collega Valente) alla fine è un provvedimento del tutto diverso da quello che ci aspettavamo, perché restringe moltissimo il perimetro di applicazione. Lì ci sono questioni annose che vanno affrontate. Se si fa un intervento legislativo, non si capisce perché viene creato un precedente che riduce lo spazio di azione, anziché alimentarlo. Tanto valeva aspettare e riflettere ancora sul punto. Poi ci sono una serie di questioni che non so se chiamare post-calamità o pre-calamità, perché purtroppo sono continuative. Mi riferisco al dramma della siccità: oggi abbiamo una prima stima della Legacoop, che parla di 4 miliardi di danni e di oltre 30.000 disoccupati nel comparto agricolo e nel comparto della pesca, a causa della siccità che sta interessando tutto il Sud d'Italia. Avevamo presentato degli emendamenti, collegandoli ai fondi FSC, che parlavano di dissesto idrogeologico, per individuare una cabina di regia che, approfittando del veicolo di questo decreto, iniziasse a dare delle risorse. Anche in quel caso ci è stato risposto che se ne parlerà

fornire strumenti aggiuntivi per il contrasto agli incendi che già si stanno manifestando, ma anche in quel caso non ci è stata data alcuna risposta. Da ultimo vorrei citare un caso che mi sta particolarmente a cuore perché è emblematico. In Sicilia nel 1990,

Questo diventa un caso emblematico. Io ho incontrato spesso, perché riguarda il mio collegio elettorale, soggetti che attendono questi rimborsi; sono soggetti molto anziani

Stato. È su questa speranza, sul ruolo delle istituzioni e sulla capacità che noi abbiamo di lenire i danni e i dolori che derivano da queste tragedie, che credo debba fondarsi il nostro intervento e l'impegno unitario di quest'Aula. esame non raggiunge questo scopo, ma, al contrario, dice alle persone che, in effetti, quando pensano di essere sole

Signora Presidente, onorevoli colleghi, con il provvedimento in discussione introduciamo disposizioni urgenti e necessarie, finalizzate a realizzare alcune specifiche esigenze emerse in sede attuativa, correlate ad eventi di Protezione civile e ricostruzione post-calamità. Occorre però premettere che la gestione dei rischi, quindi tutto ciò che è Prenotazione civile, in Italia assume un tratto particolare, perché il nostro territorio è fragile in quanto giovane: l'Italia ha solo venti milioni di anni e ciò la rende vulnerabile dal punto di vista sismico e idrogeologico. e la ricerca ambientale (ISPRA) ha censito 628.000 frane, due terzi del totale di quelle europee. Pertanto, il tema del provvedimento ha natura decisiva e lo sarà sempre più anche in relazione al famigerato cambiamento climatico e dunque a eventi estremi e ciclici.

Il nostro territorio è geologicamente giovane, sismico, esposto a frane e anche alla crisi demografica: tra il 2022 e il 2023, l'Italia ha perso circa 253.000 abitanti, l'equivalente del Municipio X di Roma, dove io risiedo, o dell'intera popolazione di Venezia. Crisi demografica, natura orografica ed eventi geologici avversi sono un *mix* che richiederebbe un'attenzione dedicata e particolare nell'ambito delle politiche del *new green perché più il suolo è abbandonato dall'uomo che se ne va, più è incolto e maggiori sono i rischi di piangere quello che è accaduto a Campi Bisenzio, in Romagna o nelle Marche. Si tratta, pertanto, di non avere un approccio ideologico e quindi facile ai temi ambientali, ma identitario e programmatico, passando dall'inseguire le emergenze a pianificare gli strumenti per prevenirle ed essere preparati adeguatamente agli eventi calamitosi. colleghi, altro che dare le colpe alle nutrie o a chicchessia. In merito agli interventi che mi hanno preceduto, vorrei chiedere intanto come mai la gestione commissariale che riguarda il terremoto del 2012 è ancora in piedi? Come mai il Governo Meloni ha stanziato 34,6 milioni per la Provincia di Ravenna e 12,2 milioni per il Comune di Ravenna e il sindaco e il Presidente della Provincia di Ravenna ne hanno utilizzato solo il 4,5 Perché molti amministratori del PD non hanno ancora utilizzato i soldi messi a disposizione dal Governo? Un giorno ce lo spiegherete, nel frattempo non ci limitiamo, con questo provvedimento, a fornire solo sostegni economici, ma rafforziamo anche le capacità amministrative degli enti locali. Viene infatti previsto il finanziamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, viene delineata chiaramente la gestione commissariale straordinaria per assicurare una risposta coordinata ed efficace. Le misure previste non solo rispondono in modo tempestivo alle emergenze che hanno colpito le nostre Regioni, ma rappresentano anche il punto di partenza per una visione strategica per il futuro, in netta contrapposizione con un approccio senza prevenzione e di solo tamponamento portato avanti in precedenza. Il nostro operato è quindi un chiaro esempio di come un Governo responsabile e attento possa fare la differenza nella vita dei cittadini e in tempo reale, quindi non aspettando il 2023 per sollecitare rimborsi riferiti ad un terremoto del 1990, quando quei rimborsi li si sarebbe potuti sollecitare tranquillamente quando si era già al Governo, quindi anche dieci anni fa. Non ci limitiamo a tamponare il disastro, ma lavoriamo per costruire una resilienza duratura, assicurando che le comunità colpite possano risollevarsi e prosperare nuovamente. Ecco perché abbiamo voluto sostenere il ruolo dell'Agenzia ItaliaMeteo, alla quale spetta l'importantissimo compito di supportare lo Stato e le Regioni nelle funzioni di protezione civile. Ma tutto questo sarebbe difficile senza risorse umane adeguate, perché l'Agenzia fino all'emanazione di questo decreto non poteva considerarsi ente di nuova istituzione e quindi semplicemente non avrebbe potuto assumere. Con questo testo diamo il via libera alle assunzioni per un ulteriore periodo di cinque anni, in modo da allargare il numero di tecnici di cui l'Agenzia potrà disporre per meglio operare. Nella seconda parte di questo testo poniamo attenzione alla sicurezza e alla protezione civile per i grandi eventi internazionali come il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Queste *kermesse* rappresentano una straordinaria opportunità per l'Italia, ma richiedono una preparazione meticolosa e un'attenzione scrupolosa alla sicurezza. Il Governo Meloni ha messo dunque in campo misure rafforzate in questo senso, dimostrando la capacità di pianificare ed organizzare con competenza e attenzione, perché abbiamo il dovere morale di agire per il bene della nostra Nazione garantendo sicurezza, sviluppo e anche, sì, prestigio internazionale. È vero che ora, nel momento in cui approviamo questo decreto, il G7 di Borgo Egnazia è concluso, ma era più che giusto prevedere risorse straordinarie per le Forze armate, per le forze di Polizia e altresì l'impiego di personale specialistico, come i reparti nucleare, che hanno consentito lo svolgimento di un evento di tale caratura in maniera impeccabile ed encomiabile. Un vertice che innanzitutto ha fatto apprezzare la Puglia, la mia terra, a livello mondiale, grazie al suo mare, al suo cibo, alla sua ospitalità e alla sua capacità di essere all'altezza organizzare eventi di questa straordinaria rilevanza e di essere lo specchio meraviglioso di questa nostra Nazione. Il *summit*, tanto per ricordarlo, sarà ritenuto importante anche in futuro perché è tra i pochi ad aver adottato una dichiarazione finale, a dimostrare innanzitutto il clima di unità di intenti, ma anche la grande capacità di Giorgia Meloni di mediare e convincere sugli impegni da portare a termine sulle sfide globali che ci investono in questo tempo difficile. E che dire del *parterre* e degli incontri? Abbiamo ospitato i vertici ONU, Banca mondiale, Fondo monetario internazionale, all'incontro hanno partecipato Papa Francesco, il presidente Zelensky, il Presidente di turno dell'Unione africana. Alcune di queste partecipazioni non erano mai state neanche ipotizzate, eppure questo Governo le ha poste sul piatto e le ha realizzate e con questo abbiamo voluto dare un altro segnale molto importante, e cioè che il G7 non deve essere uno spazio elitario chiuso, non è una realtà che deve difendersi da qualcosa o da qualcuno, ma è invece un'offerta di valori che vuole aprirsi al mondo per cercare insieme soluzioni legate allo sviluppo di tutti. A Borgo Egnazia abbiamo ribadito che non si tratta di mettere l'Occidente contro il resto del mondo, ma lavorare insieme per unire gli sforzi, per regolamentare, ad esempio, l'intelligenza artificiale, convergere sugli obiettivi per fermare le guerre e, infine, costruire un nuovo modello di sviluppo e di cooperazione con le Nazioni africane, basato su un partenariato da pari a pari perché queste possano crescere e prosperare con le risorse che possiedono e in abbondanza. la notizia della firma di Cassa depositi e prestiti e del presidente della Banca africana di sviluppo che consente il lancio del Growth and resilience Africa fund (GRAF), lo strumento finanziario dedicato all'investimento in progetti promossi da soggetti privati nel quadro dell'attuazione del Piano Mattei. La piattaforma punta ad accelerare l'attuazione di nuove iniziative promosse dal settore privato nel continente africano creando un unico punto di accesso per le opportunità di investimento e consentirà alle due istituzioni di capitalizzare fino a 400 milioni di euro in cinque anni.

Questi due ulteriori strumenti completano l'architettura finanziaria concepita a sostegno dell'attuazione del piano, rafforzando la collaborazione strategica con la Banca africana di sviluppo. insomma di un G7 ambizioso e lungimirante, e soprattutto un Piano Mattei con fondi, obiettivi, risorse, progetti e tempistiche, a differenza di chi prova ancora a definirlo come una scatola vuota senza contenuti. il decreto-legge ricostruzione il Governo Meloni non lascia soli né famiglie, né i territori, agisce sulla prevenzione, ma soprattutto dimostra di avere a cuore

che dispone che la Fondazione opera in regime di diritto privato. L'articolo 11, al comma 1, chiarisce che le attività svolte da Fondazione Milano-Cortina 2026

C'è da dire che il regime di diritto privato indica la normativa di riferimento da applicare alla gestione, ma non indica la natura del soggetto. Tutte le società pubbliche operano in regime di diritto privato, applicando il codice civile integrato da norme speciali. La principale è il testo unico sulle società a partecipazione pubblica per adattare il diritto pubblico alla funzione pubblica anche con limitazioni e obblighi diversi da quelli previsti dal codice. In definitiva le società pubbliche operano in regime di diritto privato, ma mantengono la natura pubblica. Il Governo Meloni ha tentato di dare una risposta senza modificare l'articolo 2, ma interpretandolo con la specifica che le attività della Fondazione, solo per questo e senza alcuna altra modifica legislativa, non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. La qualifica è però una cosa diversa dalla natura. I riferimenti giurisprudenziali che vengono richiamati nel provvedimento sono quelli del TAR (Piemonte 2004), quattro pareri dell'Avvocatura di Stato del 2020 e del 2021 e sentenze del Consiglio di Stato del 2018 e del 2022. Questi riferimenti giurisprudenziali sono superati però dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea recepite dalla Cassazione a sezioni unite del 2021 e del 2023.

La direttiva europea n. 24 del 2014, norma di diritto superiore, prevede che un ente sia da considerarsi pubblico se opera nell'interesse generale e se il finanziamento è pubblico. Fondazione Milano-Cortina è il comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali, che è un progetto di interesse nazionale per la realizzazione di un evento sportivo memorabile e sostenibile, che lasci positiva eredità alla nostra azione, controllato da (CONI), Regione Lombardia e Veneto, Comuni di Milano e Cortina e, dal 2022, anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle Province di Trento e Bolzano. Esso indica anche quali opere devono essere fatte, in quali luoghi e con quale cronoprogramma. Fondamentalmente quindi la natura pubblicistica della Fondazione è tale perché persegue uno scopo d'interesse generale di natura non commerciale o industriale, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia nel rispetto della Carta olimpica. Lo farebbe con denaro, membri e garanzie dello Stato e degli enti locali chiamati a ripianare alla fine l'eventuale *deficit* di bilancio dei giochi. E lo farebbe senza assunzione imprenditoriale del rischio d'impresa. Andiamo allora a vedere il bilancio della Fondazione Milano-Cortina:

premetto che la Fondazione è un ente con personalità giuridica, quindi separa il suo patrimonio da quello degli amministratori e che tale condizione è regolata dal DPR n. 361 del 2000, che all'articolo 1 stabilisce che deve possedere un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo, ossia un patrimonio minimo non definito (se non è definito, dev'essere superiore a 1). Lo statuto della Fondazione, approvato nel 2019, per recepire il principio dell'adeguatezza di quell'articolo 4, vincola 50.000 euro a garanzia dei terzi, stabilendo che, quando diminuisce o è d'importo inferiore, il consiglio d'amministrazione deve deliberare senza indugio, cioè immediatamente, quanto necessario per l'integrazione sino al suo ripristino o, in caso contrario, per la trasformazione, la fusione o lo scioglimento, cioè la cessazione di ogni attività. Allora, siamo al 2022 e abbiamo un debito (un rosso!) di 85 milioni di euro, ma il 17 gennaio 2023, prima di ufficializzare il bilancio con la perdita, questa disposizione a garanzia della presenza del patrimonio minimo è stata eliminata con una modifica dello

interpretazione autentica della norma casca in un momento in cui sono pendenti indagini a proposito della Fondazione con un'imputazione di reati diversi a seconda della natura giuridica della fondazione pubblica o privata. C'è stato il giudizio del riesame e fondamentalmente ora i capi d'imputazione sono cambiati e sono stati trasformati in modo adeguato alla nuova interpretazione della norma come ente privato. Mi chiedo se questo Governo per caso non intervenga con una falsa procedura d'urgenza per andare a incidere e condizionare il potere giudiziario: spero di aver interpretato male.

e soprattutto, almeno in una circostanza del genere, che si evitassero le solite speculazioni politiche. E invece proverò a dire in questi pochi minuti a mia disposizione perché non ci siamo trovati di fronte né all'una né all'altra cosa. Intanto, vi sono stati scarsissimo rigore e scarsissima serietà

difficile anche seguire la genesi e l'abbinamento di due provvedimenti che avrebbero dovuto avere sostanzialmente *ratio* diverse.

pochi mesi fa. In quello stesso provvedimento noi richiedevamo interventi di carattere più strutturale, che in parte sono inseriti in questo provvedimento, in maniera peraltro abbastanza confusa. Quindi, il metodo il metodo è pasticciato, come dicevo, anche perché si prova ancora una volta a rispondere - mi verrebbe da dire e del resto è nel titolo principale del provvedimento - a questa logica dell'emergenza: inseguiamo l'emergenza. Vale ovviamente per un'alluvione imprevedibile o imprevista (in gran parte imprevista, perché sappiamo che che anche quelle in parte sarebbero prevedibili, ma almeno è giustificato), sicuramente meno nel caso dei Campi Flegrei. I Campi Flegrei - com'è noto a tutti ormai, perché ne abbiamo discusso tante volte - sono una zona vulcanica enorme della città di Napoli,

case che tremano, costoni che cadono, parti di case lesionate, tanti sfollati. Stiamo parlando anche di una zona densamente popolata. Vengo ora alle critiche più di carattere politico: mi verrebbe da dire che ancora una volta il Governo perde l'occasione per dimostrarsi all'altezza della sfida che gli italiani, nostro malgrado, gli hanno delegato: il governo di questo Paese. Ho letto oggi, devo dire con non poco rammarico (non dico stupore, ma rammarico sinceramente), le dichiarazioni del ministro Musumeci nella Commissione parlamentare per le questioni regionali a proposito dei Campi Flegrei,

che puoi fare, ovviamente, e che è nelle tue mani, i cittadini e le cittadine che in questo Paese chiedono semplicemente di essere bene amministrati. *(Applausi)*. Le speculazioni politiche non servono, soprattutto quando giocate sulla pelle delle persone e non servono, perché sarebbe molto facile ricordare al ministro Musumeci - vorrei proprio usare un altro tono - che nel 2003 l'allora giunta Bassolino, con assessore all'urbanistica il nostro ex collega Marco Di Lello, aveva varato una legge, in quel caso per la zona vesuviana, che parlava già dei Campi Flegrei e diceva: attenzione, bisogna diminuire la pressione abitativa, non si può più edificare su quei territori. Ebbene, non vi sorprenderà sapere che negli anni successivi questa legge è stata ostacolata dal governo Caldoro e da tutte le forze di centrodestra che si sono susseguite e i governi, allora anche di centrodestra, non hanno mai prestato il fianco. Quindi, è troppo facile la speculazione. Io vorrei che tutti quanti insieme approfittassimo anche di di un tempo che purtroppo cambia, di una natura che purtroppo si ribella e che ci chiama tutti quanti a un senso di responsabilità maggiore di quello che dimostriamo e voi state dimostrando e che, spinti anche da questo, provassimo a esercitare un po' più di rigore e di etica della responsabilità. Capisco che è un appello che a volte rischia di cadere nel vuoto con questo Governo, ma io sono una donna molto ostinata da questo punto di vista e continuo a confidare che a un certo punto vi sia un sussulto di dignità. Ho sentito parlare

Ma dico di più. Il ministro Musumeci ha detto che il tema è quello delle risorse. Non è soltanto quello delle risorse. Con molta responsabilità, i sindaci e gli amministratori che sono stati auditi su questo provvedimento non hanno chiesto soltanto più soldi,

rispondendo quasi a una logica che sembrava sostanzialmente accentrare. Il Governo quale interesse aveva? Quello di dire: eccoci, adesso siamo arrivati. Visto che voi non siete stati capaci, ce la vediamo noi,

previsto dalla vecchia normativa. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ci ha detto che ci stanno già lavorando. Volete accentrare il potere nel nuovo commissario? Nessun problema, ma dateci almeno una norma transitoria che dica come i poteri del vecchio commissario, che era quasi in dirittura d'arrivo, passano al nuovo commissario; e spiegateci, almeno, cercate di delineare un quadro chiaro, perché così finirete solo per aggiungere confusione a un lavoro che, anche tra tante fatiche, si sta portando

che chiedevano i nostri amministratori: solo buongoverno e buona amministrazione. Vi chiedevano di non fare un ulteriore atto di speculazione sul nostro territorio, del quale non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di serietà, di rigore e di interventi che cerchino in qualche modo di fronteggiare un fenomeno che è

volta, soltanto un intervento di facciata, assolutamente speculativo e che soprattutto guarda, ancora una volta, solo agli interessi di parte e poco agli interessi degli italiani.

fra i fattori che rendono l'Italia una Nazione incredibilmente meravigliosa vi è lo sterminato patrimonio di racconti tradizionali, i quali hanno dato forma a un ricco immaginario, che varia di Regione in Regione, di città in città e di vallata in vallata. Nella mia Regione, il Friuli Venezia Giulia, una celebre storia popolare vede protagonista un terribile essere mostruoso, un orco dalle dimensioni eccezionali. Secondo la leggenda, quest'orco sarebbe stato rinchiuso nelle cavità montane della Carnia e, ogniqualvolta compie un movimento, la sua straordinaria potenza farebbe tremare la terra. Il 6 maggio 1976, pochi secondi dopo le ore 21, l'Orcolat - così viene chiamato in friulano - rase al suolo 45 Comuni e in altri 92 provocò un'innumerevole serie di danni, causando la morte di quasi mille persone in 59 secondi, 18.000 edifici distrutti, 75.000 danneggiati e lo sfollamento di più di 100.000 cittadini. L'Orcolat è ancora oggi considerata una delle più grandi tragedie che abbia mai colpito nel secolo scorso la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'intera Italia. Il 27 marzo di quest'anno il mostro è tornato a farsi sentire, questa volta con più lieve intensità e senza cagionare danni a cose o persone. Ho scelto di fare questa premessa perché - come ogni racconto fiabesco che si rispetti - anche da quello dell'Orcolat si può trarre una morale: nessun uomo, infatti, è mai andato alla ricerca del mostro per sconfiggerlo e ucciderlo, perché non ne sarebbe capace. L'essere rimane prigioniero della propria rocciosa cella, mentre la popolazione locale è consapevole che potrebbero esservi dei movimenti da parte sua anche improvvisi. Il popolo convive tutelandosi da questa eventualità com'era e dov'era, perché non è, per tante ragioni, in grado di fare altrimenti. Fenomeni sismici, anche altamente violenti, hanno afflitto e affliggono con frequenza la nostra Penisola; in ampie aree della stessa, alla sismicità è talvolta correlato il vulcanismo e costituiscono due rilevanti fonti di pericolosità naturale che, in un territorio ad alta intensità di insediamenti umani come il nostro, incrementano notevolmente il livello di rischio al quale si trova sottoposto il Paese. In aggiunta a ciò, il particolare assetto morfologico, con sovente il contributo purtroppo del fattore antropico, aumenta anche il rischio idrogeologico, rendendo l'Italia complessivamente un territorio ad alta fragilità. Con questo tipo di eventi - lo ribadisco - la convivenza è praticamente inevitabile. Tuttavia, in questo contesto assumono valore fondamentale due aspetti: la preparazione preventiva ai fenomeni e la capacità, tramite una solida organizzazione, di reazione successiva agli stessi. Sono esattamente questi due aspetti i pilastri sui quali il provvedimento di oggi si fonda. Con riguardo alla prevenzione, è necessario menzionare tutte le misure relative alla situazione emergenziale nei Campi Flegrei. Con questa disposizione viene innanzitutto istituito un commissario straordinario che, coadiuvato da una struttura di supporto di professionisti ad alto livello, resterà in carica fino al 31 dicembre 2027 e avrà ampi poteri sostitutivi in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, specialmente in materia di attuazione del PNRR e di realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica. Il commissario straordinario sarà incaricato, tra l'altro, della gestione della messa in sicurezza degli edifici ad alto rischio siti nell'area che si espande tra i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, ponendo come prioritari gli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità. Se dobbiamo farlo noi, probabilmente chi ci ha preceduto non lo ha fatto. La continuità scolastica è anche oggetto di una disposizione specifica che va a stanziare fondi per il ripristino e la riqualificazione sismica delle scuole danneggiate e sgomberate per inagibilità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio. I nostri ragazzi, dunque, sono come sempre posti al centro dell'azione di questo Governo, un Governo dei fatti: non possono essere loro le vittime dell'incuranza e della sottovalutazione del rischio che, per troppi decenni, ormai hanno caratterizzato l'operato di alcune amministrazioni, le quali si sono spesso dimenticate di risiedere in una delle zone più a rischio sia sismico che vulcanico d'Italia, se non dell'Europa intera. L'elemento preventivo è altresì valorizzato con il rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della protezione civile attraverso l'incremento del personale in organico. L'ho già detto e lo ripeto: la mia Regione è il Friuli-Venezia Giulia e, come un po' tutti i miei corregionali, provo uno smisurato sentimento di riconoscenza nei confronti della Protezione civile. Il Friuli non potrà mai dimenticare l'eccezionale supporto ricevuto dopo il sisma del 1976, coordinato dall'allora commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, il quale, fatto tesoro di tale esperienza, ebbe l'intuizione, da Ministro, di dare a tale struttura organizzativa carattere permanente. Il modello di ricostruzione di Zamberletti è stato studiato in tutto il mondo ed è pertanto nostro dovere onorare la sua eredità amministrativa, ponendo la sua creatura nelle migliori condizioni possibili per lo svolgimento della propria delicata e complessa attività. *(Applausi)*. L'incremento di personale, dunque, va in questa direzione. Colgo in quest'Aula l'occasione per porgere i migliori auguri di buon lavoro al dottor Ciciliano, Ciciliano, nuovo capo della Protezione civile nazionale. Sono certa che, grazie alla sua notevole esperienza, dimostrata anche nella realtà di Caivano, saprà ricoprire questo ruolo con efficacia e competenza. Non solo. In tema in tema di prevenzione, ci tengo a citare l'articolo 9, che permette all'Agenzia ItaliaMeteo di estendere, per un ulteriore quinquennio, l'efficacia temporale del regime speciale di reclutamento previsto dalla legge per gli enti pubblici di nuova istituzione, al fine di garantire all'ente il tempo adeguato per attivare e portare a termine tutte le procedure di assunzione e giungere così alla piena dotazione organica prevista dalla legge istitutiva. Il contributo che le scienze dell'atmosfera possono dare alla Protezione civile, in particolare attraverso le previsioni e i modelli meteorologici e climatologici, è difatti ancora troppo sottovalutato, ma è essenziale, specialmente nell'ottica di una migliore gestione dei fenomeni atmosferici violenti, nonché dei periodi di siccità che sempre più frequentemente si abbattono sulla nostra Penisola. Per quanto concerne la capacità di pronta ed efficiente reazione nella situazione post-evento, il provvedimento in discussione interviene non solo nelle succitate aree della Regione Campania, tramite i contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali divenuti inagibili a seguito del sisma del maggio scorso, ma anche con misure rivolte ai territori ai territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023 e ai Comuni dell'Abruzzo danneggiati a seguito del sisma del 2009. Nello specifico, con riguardo ai territori colpiti dalle alluvioni, la norma prevede una serie di contributi assegnabili dal commissario straordinario, del quale viene altresì prolungato il mandato, per interventi di ricostruzione privata, in particolare di beni immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi, o per l'acquisto di aree alternative o di nuovi immobili in cui delocalizzare abitazioni o attività precedentemente site in edifici gravemente danneggiati, per i quali la ricostruzione *in loco* risulta impossibile. Allo stesso tempo, è inoltre migliorata la disciplina delle verifiche a campione sugli interventi per i quali i suddetti contributi siano già stati erogati. Viene così previsto il coinvolgimento di tutti gli enti pubblici e degli organi statali aventi competenza nell'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza, per per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici. Si intende evitare, in altri termini, che i fondi pubblici stanziati per soggetti realmente necessitanti vengano deviati nelle tasche di coloro che, sulle tragedie e sulle emergenze, sono soliti lucrare senza dignità, come si è visto anche nel recente passato, in numerose altre occasioni. Ogni riferimento alla crisi pandemica e al superbonus 110 è puramente voluto. *(Applausi)*. Inoltre, mi preme menzionare che, relativamente ai Comuni in Abruzzo danneggiati dal sisma del 2009, con un'interpretazione autentica l'articolo 7 chiarisce che possono rientrare dietro condizioni anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, relativamente ai territori abruzzesi colpiti dal sisma. Questa misura contribuisce all'ingresso di un nuovo flusso di risorse destinate a quei Comuni che a fatica, ma con tenacia, stanno rimettendosi in piedi dopo essere stati piegati da quel terribile avvenimento, che ancora oggi risiede indimenticato nella memoria di tutti noi. Ho cominciato il mio intervento con l'immagine di un orco che, secondo la leggenda, vivrebbe rinchiuso tra i monti del Friuli. La verità è che ogni territorio della nostra straordinaria Nazione si trova a dover convivere, purtroppo, con un mostro che in diverse modalità affligge la popolazione locale, anche tramite certe amministrazioni. Ciò che è necessario è farsi trovare più pronti possibile nel momento in cui l'evento accadrà e, in seguito a ciò, avere a disposizione una struttura di supporto statale, quando sarà il momento di ripartire e ricostruire. Questo ci ha insegnato il terremoto in Friuli, nei quindici anni necessari per la completa ricostruzione. E ai polemici interventi di questi giorni, anche durante l'esame in Commissione,

raccolta dall'allora giovanissimo Gianni Minà nelle ore successive alla tragedia del 1976 a Casasola di Majano: a cosa serve piangere? Qui bisogna ricostruire e non piangere.

il testo che oggi ci accingiamo a discutere e di cui domani voteremo gli emendamenti segna ancora una volta la differenza - ne è proprio la prova pratica e tangibile - tra la narrazione questo Governo continua a fare di sé, della sua attività, dei suoi programmi, dei risultati che sostiene di raggiungere, e la realtà dei fatti. Se non ci fosse una differenza fra ciò che il Governo narra di riuscire a fare e di avere fatto

che nasceva per introdurre misure per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento dei grandi eventi internazionali, non ci sarebbe stato bisogno di emendare il testo a cura della maggioranza e dello stesso relatore, aggiungere un corpo ulteriore di norme riguardanti i Campi Flegrei, per i quali il Governo aveva emanato un decreto-legge appena qualche mese fa.

sentito parlare di amministratori locali che non sono stati in grado di arginare gli interventi urbanistici, di evitare che si creassero le condizioni che poi hanno dato luogo al dramma conseguente a una calamità naturale.

la buonafede, o almeno un'onestà intellettuale. Ci provo ma, leggendo questo ennesimo decreto-legge, mi rendo conto che c'è ben poca onestà intellettuale in questi provvedimenti. Dico ciò perché perché leggo un testo che parla di ricostruzione post-calamità e interventi di protezione civile e comprendo anche dalle parole di chi mi ha preceduto, anche dei senatori e dei colleghi della maggioranza, che si vuole dotare la Protezione civile di risorse, che si vuole avere un approccio anche programmatico e strategico; poi, però, nel testo in esame non trovo un articolo, una disposizione che si occupi di programmazione, prevenzione e monitoraggio. E parlo non di monitoraggio delle aree già colpite da sisma, da bradisismo e da alluvioni, ma di prevenzione sul territorio nazionale. Infatti, che l'Italia sia un territorio fragile ormai è una verità assodata, sulla quale non c'è neanche bisogno di andarsi a dilungare, tant'è vero che negli interventi che mi hanno preceduto abbiamo avuto memoria e testimonianza di terremoti

si fanno interventi soltanto emergenziali che si limitano a mettere delle somme, per esempio, per rifondere l'acquisto del vano cucina per le zone alluvionate del 2023, prevedendo un importo di 3.200 euro fino a un massimo di 6.000 euro per recuperare gli arredi degli appartamenti degli appartamenti colpiti dal fango. Si prevedono delle misure emergenziali per gli sfollati che hanno dovuto abbandonare la propria casa e solo adesso, dopo sei mesi, ci si ricorda di quando li abbiamo buttati fuori da casa. di vista, è un grande interprete dell'emergenza sempre più devastante: prima vara un programma di abbandono delle case

Vedete, quando manca il monitoraggio; quando manca un piano di valutazione della vulnerabilità sismica, che può essere fatto non solo ed esclusivamente per le zone dei Campi Flegrei, ma per tutta Italia; quando ci si dimentica di inserirlo in un testo del genere, allora davvero la domanda è chiara: stiamo aspettando un altro evento per fare questo genere di interventi anche nella prossima zona che sarà colpita da qualche sisma naturale? Davvero dobbiamo aspettare e ricorrere alla decretazione d'urgenza sempre con questo scopo? Eppure, ricordo che era stata creata un'unità di missione, che erano state previste proprio dal Governo Renzi le strutture per contrastare il dissesto idrogeologico e la vulnerabilità del territorio: somme che sono state immediatamente eliminate, finalità che non sono state più perseguite, obiettivi che non interessano a nessuno, come non interessano a questo a questo Ministro. Mi dispiace che non sia in Aula, questa sera, il ministro Musumeci, perché sarebbe stato bene che ascoltasse quello che l'Assemblea aveva da dirgli. E mi dispiace che in questo decreto-legge non sia previsto neanche un euro di risorse per il contrasto agli incendi,

travolti abitazioni, coltivazioni e animali e le persone hanno perso anni di sacrifici. In quell'occasione, appena un anno fa, il ministro Musumeci venne in quest'Aula - me lo ricordo molto bene lamentandosi del fatto che era difficile reperire i Canadair per un problema di monopolio di fatto della società che li costruisce e per la difficoltà del Governo ad acquistare aeromobili vitali ai fini del contrasto degli incendi. È passato un anno e non mi pare sia cambiato nulla. E, quindi, quella che era l'emergenza incendi continua a essere tale e il decreto-legge che viene varato proprio con la finalità di potenziare la Protezione civile, e quindi per fronteggiare questo tipo di interventi,

Abbiamo, al solito, una visione centralista che vuole accentrare i poteri e, quindi, decide di istituire l'ennesimo commissario straordinario anche per i Campi Flegrei, che si sostituisce agli amministratori locali e alla Regione Campania; che con ampi poteri dovrebbe poter risolvere entro dicembre 2027 ogni problematica relativa alla zona,

che dovrebbe dimostrare sostanzialmente all'opinione pubblica che basta l'uomo capace al comando per risolvere le inefficienze dell'amministrazione di turno che si deve colpevolizzare. È evidente che questo è un attacco diretto all'amministrazione della Regione Campania, che deve essere fatta passare come l'amministrazione che non è stata in grado di fare nulla. *(Applausi)*. Non mi stupiscono le parole del ministro Musumeci nell'audizione di stamattina sostanza, ha addossato la responsabilità della situazione alle amministrazioni locali che non hanno impedito l'urbanizzazione e l'eccesso di edificazione, che non hanno vigilato sui territori. Sa perché non mi stupiscono, signora Presidente? Il ministro Musumeci, già Presidente della Regione siciliana, è quello che, quando era Presidente della Regione siciliana, ha perso tutti i fondi per l'emergenza idrica tutti i fondi per l'emergenza idrica *(Applausi)* e adesso si permette di rimproverare il presidente Schifani, additandogli ogni responsabilità relativa alla mancata possibilità di intervenire sull'emergenza idrica. Questo è il Ministro Musumeci, che avrei avuto il piacere di vedere in Aula almeno per sapere se, di fronte ai fatti che gli possiamo contestare con chiarezza perché riscontrabili nella loro oggettiva esistenza, avrebbe avuto almeno la decenza di dire che la colpa non è degli amministratori locali. Questi ultimi fronteggiano difficoltà

spesso assumendosi responsabilità che nessuno al posto loro si prenderebbe. Certamente, giammai. È un Ministro che siede a Roma e finge di dimenticare quello che ha fatto quando era Presidente della Regione siciliana.

di delusione, di preoccupazione e anche con disagio rispetto al modo in cui sono state gestite la discussione e l'approvazione degli emendamenti in Commissione riguardanti la ricostruzione, la protezione civile, i grandi eventi e i Campi Flegrei. Sebbene questa volta ci sia stato un minimo di discussione, l'impressione generale è che ancora una volta ci troviamo di fronte a un processo in cui mancano profondità, lungimiranza e trasparenza. È positivo che siano stati invitati e ascoltati esperti in materia, professionisti e rappresentanti degli enti locali, che hanno dedicato tempo e competenze per analizzare il decreto-legge e fornire contributi significativi. Questo non può essere sufficiente, però, se le decisioni finali non tengono conto dei dati emersi, ma si rivelano essere sempre già predefinite e precostruite, riducendo il nostro ruolo di senatrici e senatori, e anche il vostro di maggioranza, a quello di mere comparse in un copione prestabilito. Il dispendio di risorse e il coinvolgimento di personale qualificato sono importanti, ma sono vanificati se l'*iter* legislativo si conclude con la solita messa in scena in cui le scelte non risultano essere realmente influenzate dai dati scientifici e dalle analisi emerse. Il vostro approccio e il vostro modo di operare - colleghe e colleghi della maggioranza - non permettono di lavorare e legiferare seriamente con coscienza e anche trasversalmente per il bene collettivo, per risolvere concretamente i problemi dell'Italia, la quale si sta allontanando sfiduciata dalla politica, tanto che per otto italiani su dieci essa non rappresenta i cittadini. Di questo passo il sistema Italia andrà a sbattere, ma sembra poco importare alla maggioranza. È questo quello che sta succedendo. Il Governo sta andando avanti imperterrito e sordo ai veri problemi che stanno attanagliando il nostro Paese: salute, lavoro, cambiamento climatico. È sordo anche di fronte alle tante istanze che ci arrivano quotidianamente dalla società civile, dalle comunità locali, dalle imprese, preferendo spaccare l'Italia invece che unirla. Sempre più lontano dalle realtà è diventato un miraggio discutere qui di soluzioni serie che abbiano un filo di senso logico rispetto alle sfide e alle criticità da affrontare nel nostro presente. Il Il Governo e voi della maggioranza sempre più compulsivi continuate imperterriti a operare in un atteggiamento di ostinata chiusura; armati di paraocchi, proseguite dritti su una strada vecchia e inefficace, ignorando le necessità di adottare approcci moderni e innovativi. La gravità di alcuni problemi che stanno tormentando l'Italia e che ogni giorno si acuiscono per mancanza di azioni concrete - come rilevato anche prima dai miei colleghi - dovrebbe farci sobbalzare dalla sedia. invece a votare la conversione di questo ennesimo decreto-legge *patchwork* in materia di ricostruzione, protezione civile, grandi eventi, Campi Flegrei, che non fornisce una risposta adeguata ai problemi che vivono quotidianamente le nostre comunità e non indica la corretta strada da intraprendere per garantire un futuro sempre più giusto, equo e ambientalmente sostenibile. La prima obiezione che voglio avanzare è per me la più chiara e inequivocabile. Dov'è possibile, è assolutamente necessario evitare di consumare di nuovo il suolo. Solo per memoria: quello del consumo netto zero da raggiungere entro il 2050 è un obiettivo europeo a cui abbiamo il dovere di ispirarci, e non perché è l'Europa che ce lo chiede, ma perché dobbiamo contenere in tutti i modi i danni devastanti che il cambiamento climatico sta causando all'Italia. La sistemazione degli sfollati per eventi alluvionali, per esempio, dovrebbe avvenire prioritariamente utilizzando edifici già esistenti da efficientare o che hanno perso la loro funzione originaria. Una miriade di strutture dismesse potrebbe tornare a nuova vita, offrendo solidarietà solidarietà umana, riparo e speranza a chi ne ha bisogno e si trova in un momento di drammatica difficoltà. Lo Stato dovrebbe ristrutturare quelle strutture con fondi adeguati, mettendo in tal modo in sicurezza il nostro prezioso patrimonio. La seconda osservazione riguarda i nostri corsi d'acqua. L'Unione europea ci sollecita e ci raccomanda costantemente, attraverso la normativa comunitaria, di rinaturalizzare gli ambiti fluviali, evitando ulteriore cementificazione degli alberi e delle scogliere. Bisogna individuare con urgenza le aree idonee per gestire adeguatamente le possibili e sempre più frequenti esondazioni dei corsi d'acqua e proteggere le comunità locali da potenziali e futuri disastri che stanno già provocando danni incalcolabili. È da inizio legislatura che noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo di svolgere urgentemente la manutenzione della rete idrica italiana, un vero colabrodo, che disperde acqua fino al 45 quasi la metà, e lo sappiamo tutti. Bisogna impostare un serio piano strutturale e investire nella prevenzione, anziché parlare di "post", e smetterla di agire e reagire solo in emergenza, con i classici decreti siccità o alluvioni. Se non l'avete capito in due anni, con un'Italia in preda agli effetti devastanti del cambiamento climatico, mi chiedo cosa debba succedere ancora per farvi cambiare rotta. Per quanto riguarda invece l'articolo 11, relativo ai grandi eventi, esprimo la mia profonda preoccupazione per la situazione critica che sta coinvolgendo la Fondazione Milano-Cortina 2026. Lo scontro tra il Governo e la procura di Milano ha raggiunto un livello preoccupante. La magistratura definisce di gravità inaudita il decreto-legge dell'Esecutivo approvato un mese fa, che qualifica la Fondazione come ente privato invece che pubblico, rendendo più difficile l'accertamento delle irregolarità e del perseguimento delle accuse di corruzione e turbativa d'asta in corso. Tale provvedimento, secondo la procura, potrebbe rappresentare un tentativo di bloccare le indagini. Le intercettazioni e i documenti acquisiti dimostrano che la Fondazione opera effettivamente come un ente pubblico, nonostante la sua qualificazione legale di ente privato, e ricordo che le Regioni, le Province autonome e le aziende partecipate, come la Rete ferroviaria italiana e l'ENI, sono tra i principali finanziatori. Questo è un fatto di gravità inaudita, che solleva ulteriori preoccupazioni riguardo la trasparenza e la gestione dei fondi pubblici. L'inchiesta ha infatti evidenziato potenziali irregolarità negli appalti e nelle assunzioni, con sospetti di corruzione che sembra coinvolgano anche la nuova gestione dell'ente. È evidente che la Fondazione Milano-Cortina 2026 debba operare con totale trasparenza, rispettando le norme del diritto pubblico e garantendo una gestione onesta e responsabile dei fondi, a beneficio di tutte le comunità coinvolte. Questa controversia si aggiunge poi alla già criticata e scellerata gestione delle infrastrutture previste per i Giochi invernali e dei fondi per la costosa costruzione della pista da bob a Cortina, che ci sta già causando danni di immagine e di affidabilità a livello internazionale. E mentre il Governo italiano, sovranista e campanilista, si è intestardito, a spese dei contribuenti italiani, a voler svolgere le gare di bob, skeleton e slittino all'interno dei confini veneti, la Francia, a cui sono stati assegnati i Giochi olimpici e paralimpici invernali nel 2030, ha deciso di sconfinare, chiedendo a Torino di utilizzare l'impianto Oval per le gare di pattinaggio. In tal modo, i francesi spenderanno sette o otto volte in meno rispetto all'Italia, la quale, navigando nell'oro, ha già sforato il tetto dei 3,6 miliardi per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026. Furbo e intelligente il Governo a non ascoltare gli appelli per svolgere le gare di bob a Saint Moritz o Innsbruck e a voler stravolgere ambiente e paesaggio di un gioiello delle Dolomiti qual è Cortina, e questo per interessi di pochi e non per quelli delle comunità del territorio. Colleghe e colleghi, è nostro dovere gestire in modo oculato le finanze del nostro Paese. È nostro dovere lasciare in eredità alle presenti e future generazioni una Terra e un Paese più in salute, più sostenibile e vivibile per le nostre comunità e per tutto il nostro territorio. Ricordiamolo, ricordiamocelo e ricordatevelo.

Noi, come MoVimento 5 Stelle, avevamo già evidenziato quelle che erano le anomalie nel primo provvedimento e avevamo chiesto di più e meglio. Ci eravamo allora astenuti dal voto sul provvedimento, perché il faro acceso dal Governo su

eventi il cui culmine è stato il 20 maggio, con una scossa di 4.4 gradi che ha arrecato scompiglio all'interno di quella popolazione, scompiglio tale da far saltare anche quello che era il piano di evacuazione.

e l'attenzione di tutti i cittadini italiani, visto che interviene in situazioni particolari e anche in condizioni precarie in termini di risorse, durante le audizioni, proprio in merito ai Campi Flegrei, abbiamo audito il Capo della struttura della Protezione civile,

in Commissione e abbiamo sentito i sindaci, i funzionari, persone che vivono il territorio e hanno operato sul territorio. Qui faccio seguito anche a quanto diceva la collega Valente: sono state proposte delle variazioni anche a costo zero, quel caso, durante la nostra attività emendativa, ci siamo sentiti rispondere picche. Abbiamo chiesto che il nuovo commissario non andasse in sovrapposizione con le attività già in corso

All'atto della nomina del nuovo commissario decade la funzione del vecchio, per cui abbiamo chiesto una deroga per quindici giorni, o almeno che entro quindici giorni dalla nomina del nuovo commissario venissero quantomeno prese in atto quelle quelle attività per poi permettere di completarle e non aspettare il continuo funzionamento. Lì c'è stato risposto picche. Abbiamo chiesto poi degli interventi economici. Il mantra è stato: il MEF Ogni volta che ci sono stati bocciati gli emendamenti e chiedevamo quale fosse la motivazione, la risposta era: lo dice il MEF. Ma su elementi che riguardano la vita dei cittadini, il MEF dovrebbe fare ben poco. Dovrebbe rispondere alle esigenze dei cittadini, così come dovrebbe fare il Governo. I soldi poi si trovano.

ad accusare i cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei, perché hanno costruito ed hanno costruito male. In genere, davanti a eventi calamitosi, si mostra solidarietà. In questo caso, invece, si va in giro a denigrare un intero popolo. Questo, in realtà, non dovrebbe rientrare nelle funzioni di un Ministro, che dovrebbe tutelare i cittadini sempre e comunque. Abbiamo chiesto un finanziamento maggiore per le scuole, chiesto un finanziamento maggiore per le scuole, perché noi sappiamo che le scuole già di per sé hanno dei vizi, vizi di collaudo o meno. Quindi, soprattutto in un caso del genere, in territori dove potrebbero intervenire - il bradisismo non si è certo fermato - abbiamo chiesto un impegno maggiore. MEF ha detto che non ci sono i soldi. Ma se non si aiutano le scuole e i futuri cittadini? Ci lamentiamo di zero nascite e poi, invece, non andiamo a tutelare chi al momento sta crescendo e il posto dove la sicurezza deve essere applicata in modo maggiore.

che il Comune ed il Governo devono intervenire con delle cifre, con un sussidio, abbiamo chiesto di dare magari un aiuto a chi mette a disposizione la propria casa.

Bisogna intervenire sulla pianificazione, sul controllo della sismicità degli immobili, siano essi pubblici o privati. Ebbene, dopo otto mesi, questo piano non è ancora stato operato.

il dramma è avvenuto. Quando poi il dramma avviene, infatti, il cittadino scende per strada e la disperazione dei cittadini sarà sempre e comunque a carico dello Stato, perché non può essere certo abbandonata a sé stessa una cittadinanza intera. Quindi, con questo provvedimento, che riprende solo in parte quello che avevamo chiesto e per cui avevamo dato fiducia, con un'astensione, al decreto del 2023, ritroviamo che poco è stato fatto, a volte anche in modo confusionario. Penso al il Governo ha messo a disposizione 184 milioni per operare sugli immobili che avevano subito dei danni classificabili come alti e medio alti. Questa classificazione, effettuata dalla regione Campania, ha valutato quasi 1,2 miliardi, dando vari livelli di classificazione, fino a arrivare ad alto

inseriamo all'interno di questa classificazione anche gli interventi classificati con importanza media; che ci sia o meno da aggiungere un'ulteriore somma, quantomeno copriamo una parte di quei lavori classificata all'interno di di quei lavori classificata all'interno di questo piano. Ebbene, anche lì c'è stato detto che il commissario spenderà quella cifra in eccedenza, magari chiedendo un controllo al Governo. Abbiamo

vi è stata la maggiore delle scosse sismiche che hanno colpito quel territorio, e la data odierna, a fine di luglio,

di rilascio di nuovi titoli edilizi abilitativi per edifici a uso abitativo o addirittura impone alla Regione Campania di presentare un piano di riqualificazione alla Presidenza del Consiglio, nella persona del responsabile della Protezione civile. civile. Purtroppo, siamo nuovamente a dover trattare del contenuto di atti urgenti in materia di stati emergenziali e di disastri che avvengono sul territorio, ci dobbiamo contemporaneamente interessare di quelli che non sono veramente prevedibili e che possono colpire indifferentemente in tutte le parti del territorio come ad esempio le alluvioni (come le tante che hanno colpito i nostri territori), e di quelli che invece sono probabilisticamente più individuabili per particolari

delle linee operative che si quantificano in misure economiche che vengono circoscritte, ad esempio per quanto riguarda l'alluvione in Emilia Romagna, in Emilia Romagna, a contributi che vanno a favore dei cittadini per i danni che si sono verificati all'interno dell'abitazione. E anche per quanto riguarda i Campi Flegrei, perché si circoscrivono gli edifici edifici che non sono più idonei ad ospitare le famiglie e si individuano per metro quadro, in base anche al peso delle ristrutturazioni che interesseranno quegli edifici. È chiaro che dobbiamo intervenire in via d'urgenza per tamponare delle necessità che si sono purtroppo ritrovate dopo anni di sprechi e di inefficienze. Ma non dobbiamo soltanto dare delle colpe; ci dobbiamo anche rendere conto che oggi le coscienze e quindi la percezione dei pericoli sono sicuramente amplificate e migliorate, grazie alla molteplicità di esperienze che abbiamo acquisito, grazie ai numerosi strumenti che abbiamo a disposizione per poterli prevedere e grazie a un complesso sistema di volontariato che si occupa di formare i cittadini alle reazioni che bisogna avere in situazioni emergenziali. Il collega ricordava prima il caso della fuga in auto di cittadini coinvolti in una situazione di

alla struttura della Protezione civile - quella ramificazione territoriale di migliaia di volontari che quotidianamente assistono e prestano il loro gratuito intervento di fronte a queste In Emilia-Romagna e in tante altre località abbiamo assistito, soprattutto da parte a una dimostrazione di altruismo che non è facilmente individuabile in altre situazioni, visto che ci lamentiamo spesso, purtroppo, del comportamento a volte non troppo corretto di molti di loro. Noi della Lega, già nel programma elettorale del 2022, abbiamo sottolineato quanto sia importante l'istituzione di un servizio obbligatorio nell'ambito giovanile, che permetta ai giovani di svolgere in favore della comunità di cui fanno parte e di cui devono essere protagonisti, attività utili a formarsi, ad acquisire delle competenze e dare supporto alle popolazioni che purtroppo si ritrovano improvvisamente ad affrontare disastri, lutti e innumerevoli danni materiali. Penso, in questo senso, anche alla mia Toscana, che nel novembre 2023 ha subito, nell'area fiorentina di Campi Bisenzio,

oggi, con la coscienza, con le normative e con un senso civico ben diverso da quello del passato e degli amministratori che quei territori hanno amministrato, quegli errori non sarebbero ripetuti. Ci dobbiamo quindi concentrare

le nostre risorse sono destinate dieci volte di più alla situazione emergenziale che non a quella preventiva. E quella preventiva non può che nascere con il supporto degli amministratori locali. È necessario formare amministratori in grado di prevenire e in grado di intervenire senza la paura di avere, come primario interesse, quello di conseguenze elettorali che, molto comprensibilmente, possono essere una risposta a dei fastidi che a volte arrechiamo ai cittadini, quando dobbiamo loro rappresentare a quali pericoli possono essere esposti, non per colpa loro, ma per colpe che derivano da scelte che sono state fatte nel passato. nel passato. Come dicevo, il miglioramento della gestione dell'emergenza non può che riguardare anche scelte operative che questo Governo, in maniera

Mi spiace aver sentito prima delle parole di senso contrario, perché molti amministratori locali hanno riconosciuto che la realizzazione di opere che questi commissari straordinari hanno permesso di veder concretizzate sui territori colpiti da queste tragedie avrebbero richiesto anni, se fossero state pianificate e concluse attraverso dei procedimenti ordinari.

che, diversamente da quanto ci dimostra la praticità, ad oggi possono essere realizzati solo grazie all'ausilio di deroghe normative, grazie ai molti commissari straordinari che - guarda caso - sono dei generali dell'esercito, sono figure probabilmente in grado di gestire non tanto l'emergenza, ma anche l'esecuzione degli ordini impartiti. Noi siamo quindi anche orgogliosi di averne valorizzato l'immagine, attraverso quella figura figura del generale che abbiamo voluto nelle nostre liste. Riteniamo infatti questo sia il sintomo e anche l'indice di una parte della pubblica amministrazione che riesce a rendersi assolutamente utile ed orgogliosa

questa grande realtà che serve tutti i cittadini. fa riferimento a disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, è, come sempre, interessante sul piano mediatico, per la vostra capacità di fare propaganda nel Paese e in quest'Aula,

Basta questo per dimostrare il senso e il ruolo che questa maggioranza e questo Governo intendono affidare al Parlamento, perché siamo in prima lettura, a dieci giorni dalla potenziale decadenza del decreto-legge e ancora noi non conosciamo gli orientamenti del Governo per l'Assemblea. Lo stato confusionale della maggioranza e dell'intero Governo è evidente. Mi dispiace che in Aula non ci sia il ministro Musumeci e che anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento si sia allontanato, ma diciamoci con grande chiarezza che dopo il passaggio in Commissione, dopo che anche le opposizioni hanno presentato emendamenti comuni per cercare di uscire dalla dialettica della contrapposizione preventiva, che per noi è sbagliata quando si parla di ricostruzione e di interesse generale, le risposte della maggioranza sono state delle arrampicate sugli specchi, precarie, anche senza numeri, senza relazioni tecniche, con grande improvvisazione e con tanta precarietà. Dunque, se fossimo onesti, dovremmo cambiare titolo al decreto-legge decreto-legge e dire che stiamo parlando di disposizioni urgenti per rallentare la ricostruzione e per tradire gli impegni assunti dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con il testo in discussione stiamo riproponendo e state riproponendo una ricostruzione fai da te. Colleghi, non dobbiamo dimenticare che siete stati abili, a pochi giorni dall'alluvione, nelle sfilate, nelle promesse. Sarebbe da parte vostra più onesto affermare da subito che non ci sono le risorse, che avete scelto altre priorità e questo è il motivo per il quale non ci sono le risorse, perché per altre priorità le risorse le avete individuate. Ma questi cittadini emiliano-romagnoli, toscani, marchigiani sono stati di fatto presi in giro dalle promesse fatte non dalla terribile opposizione,

il riconoscimento del 100 per cento dei danni come obiettivo di questo Governo e la presidente Ursula von der Leyen aveva garantito l'impegno dell'Europa anche a individuare le procedure necessarie per non lasciare da sole le famiglie e le imprese. imprese. Colleghi, credo che siamo in presenza di un Governo in fuga, che è fuggito dalla ricostruzione, fugge dalle responsabilità, tradisce le promesse, che - attenzione - sono promesse fatte dalle cariche istituzionali. Per noi, la Presidente del Consiglio è la Presidente del Consiglio dei ministri del Governo che appartiene a tutti noi, al Paese intero, non è il capo di un partito, è il Presidente del Consiglio dei ministri che ha preso un impegno in quel territorio per la ricostruzione. Se non siete nemmeno capaci, con il Governo, che è una vostra responsabilità, di mantenere e sovraintendere alle relazioni con le istituzioni, vi faccio una domanda molto semplice: ma perché il ministro Musumeci o la presidente del Consiglio Giorgia Meloni o il sottosegretario Mantovano non convocano la cabina di regia per definire gli obiettivi di questa ricostruzione? Compito del Governo non è quello di scaricare le responsabilità ai sindaci, ma quello di garantire che la ricostruzione avvenga sul principio della leale collaborazione tra tutte le istituzioni, perché siamo in presenza di un danno grave nei confronti delle famiglie e delle imprese. Quando di mezzo c'è una calamità, non si gioca allo scontro politico, ma si affrontano le problematiche che le calamità producono nel nostro Paese. *(Applausi)*. con grande franchezza, senza voler essere frainteso: perché non si convoca questa cabina di regia e si continua a scaricare la sindaci? Lo dico rivolgendomi alla Presidente e, per suo tramite, ai colleghi di Fratelli d'Italia: l'iniziativa che avete adottato in queste ore e in questi giorni, finalizzata a dire che i sindaci sono pieni di risorse e non sanno utilizzarle, è perfino al limite della decenza, perché dovreste sapere e dovremmo sapere tutti che i sindaci non hanno potere legislativo, ma applicano le regole che questo Parlamento ha approvato e che peraltro noi non abbiamo condiviso.

a procedere in maniera strutturale, perché non si può continuare ad agire solo sulle risorse di somma urgenza e con le procedure di somma urgenza, cioè - per farmi capire - ricostruendo le strade sulle frane, ripristinando i danni degli edifici ovunque essi siano, anche se sono collocati nelle aree ad altissimo

e lo dico a un Governo che dovrebbe, prima di tutto, cambiare rotta rispetto alla negazione dei cambiamenti climatici e al ritardo nella presentazione di un piano per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Non si esce da questa situazione senza reintrodurre la parola "prevenzione". Occorre un piano strutturale per adattare, ad esempio, i reticoli idrografici dentro le conseguenze che questi cambiamenti climatici apportano. Siete al Governo da due anni e non si può continuare ad usare la retorica dell'individuare nel passato i colpevoli o addirittura di cercare uno scontro tra le istituzioni, perché le istituzioni sono di tutti

i danni più rilevanti e più evidenti sono quelli sui beni mobili, quando parliamo di famiglie. Ora mettere un tetto di 6.000 euro sui beni mobili è una presa in giro, qualcosa di precario che tradisce la promessa. A differenza di un terremoto che di fatto genera problemi strutturali agli edifici, quando una casa non crolla, i beni mobili sono al sicuro. La ricostruzione di un terremoto avviene dunque sui beni immobili. Un'alluvione che mette sott'acqua il piano interrato, il primo piano e in alcune città addirittura il secondo piano dell'edificio, crea danni ai beni mobili che non si possono quantificare in massimo 6.000 euro. Perché così si tradiscono le promesse, gli impegni e gli indennizzi che il vostro Governo ha promesso a quel territorio. Cade così la credibilità del Governo e delle intere istituzioni. E voi avete determinato uno scontro politico per gestire questa alluvione, soprattutto in una Regione laboriosa come l'Emilia-Romagna, capace di rimboccarsi le maniche.

in percentuale molto alta al PIL nazionale. Noi vi avevamo presentato proposte utili per una migliore gestione commissariale dell'evento traumatico che non dobbiamo mai dimenticare essere stato una calamità grande, tra le prime tre al mondo nel 2022. mondo nel 2022. Perché si vuole determinare uno scontro politico a tutti i costi? Perché volete insistere in uno scontro tra istituzioni? Perché non si prova a ricostruire una corretta relazione tra le istituzioni per dire la verità ai cittadini e alle imprese? la stessa cosa per il comparto agricolo. Sappiamo bene quanto pesi la produzione lorda vendibile in quelle terre per l'*export* nazionale di quel comparto. Vi avevamo semplicemente chiesto di mantenere gli impegni. Vi abbiamo proposto di mettere il commissario

Perché dobbiamo abituarci a riprogettare il contrasto al dissesto idrogeologico. Abbiamo bisogno di interventi strutturali. Nel ringraziare il dottor Curcio e nell'augurare al nuovo al nuovo direttore Fabio Ciciliano i migliori auguri di buon lavoro, voglio solo dire che il nostro auspicio è sempre che il Governo cambi strada, scelga la responsabilità al posto della propaganda per servire le istituzioni anziché usarle solo ed esclusivamente per ragionare per ragionare sul consenso. In ballo c'è la credibilità del Paese e la capacità di un territorio di produrre qualità del lavoro e sviluppo economico.

cose fuori luogo. Non ci hanno visti arrivare oppure ci hanno visti arrivare e non si sono resi conto. Non hanno nemmeno letto quello che abbiamo fatto e ciò mi preoccupa. Hanno detto che la maggioranza non ha preso atto dei cambiamenti climatici. Gli è sfuggito il PNAC. Forse ancora non avete presente che questo Governo il 23 dicembre 2023 ha approvato il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Vi ricordo che era stato presentato dal precedente Governo nel

non avrebbero fatto l'intervento che ho sentito da chi mi ha preceduto. Il PNAC consiste in 361 linee guida che individuano tutti i criteri che dobbiamo adottare per diminuire il rischio idrogeologico e per fare tutte le pianificazioni a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale affinché i nuovi sistemi ambientali, economici e sociali si adattino ai nuovi cambiamenti climatici. L'abbiamo adottato. Poi ho sentito parlare di interventi non fatti per il dissesto idrogeologico, per cui il Governo deve intervenire assolutamente. Ricordo che

alla riqualificazione del territorio per abbattere il rischio idrogeologico. Non sono arrivati, abbiamo dato la proroga al 30 aprile, ma niente; al 30 giugno, sapete quante Regioni avevano mandato i progetti? Sei. Sei. È quindi una responsabilità non solo del Governo, ma anche delle Regioni e degli enti locali: forse dobbiamo iniziare a evidenziarla, affinché poi tutto proceda nel modo giusto. Entrando nel merito, come ho detto, il ringraziamento va alla relatrice, ma sicuramente anche a questo Governo, al presidente del Consiglio Meloni, al ministro Musumeci e a tutti i Dicasteri che hanno operato per far sì che questo provvedimento diventasse quello che è oggi, perché al suo interno lanciamo due messaggi fondamentali. Anche qui, ho sentito dire che non lo facciamo, alla gestione dell'emergenza immediata: ma quello che facciamo con i nostri provvedimenti però è finalmente andare a lavorare sulla prevenzione. Noi preveniamo, cerchiamo di capire quali sono le azioni strutturali da fare sui territori al fine non solo di mitigare, ma anche ridurre il rischio morfologico, idrogeologico e anche sismico. In sintesi, vogliamo fare una programmazione vera e propria degli interventi da adottare nei nostri territori, perché fino ad oggi abbiamo invece fatto la triste conta dei danni e delle vittime, e questo purtroppo è palese agli occhi di tutti. Di interventi strutturali ne sono stati fatti ben pochi,

Mi preme evidenziare che in questi due anni il Governo italiano ha dimostrato un impegno senza precedenti nel rafforzare le misure di prevenzione e programmazione, il tutto al fine di garantire sicurezza per i cittadini e soprattutto per la resilienza delle nostre comunità. un percorso portato avanti dal ministro Musumeci, che continua a lavorare per rendere la nostra Protezione civile sempre più snella e in grado di reagire agli eventi. È stato lo stesso Ministro, in occasione della nomina del nuovo capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, a cui vanno tutti i nostri auguri di buon lavoro, a tracciare la rotta, potenziando la prevenzione e la riqualificazione delle emergenze e soprattutto accorciando i tempi per quanto riguarda le pratiche da portare all'interno degli uffici comunali, provinciali, regionali e nazionali, al fine di ottenere i famosi nulla osta in maniera rapida. L'aumento degli eventi meteorologici, come ho detto prima, è ben chiaro a questo Governo: detto fatto, l'ha tradotto adottando il PNAC. È un approccio proattivo, una novità rispetto al passato, e rappresenta una svolta fondamentale. Naturalmente, il concetto di prevenzione non è qualcosa che deve chiamare in causa solo il Governo, ma anche tutti gli altri enti, dalle Regioni alle Province, ai Comuni, ma anche ai cittadini, ai cittadini, che devono essere partecipi di questo nuovo modo di operare, perché poi sono loro, con le loro azioni, che riusciranno a conservare l'ecosistema e soprattutto il patrimonio ambientale. Come spiegato anche dal relatore, in questo provvedimento c'è tutto quanto serve per delimitare cornici operative sempre più stringenti per la vera ripartenza dei territori colpiti, dall'importanza di garantire concreti contributi ai soggetti privati colpiti dalle calamità alle misure per accelerare i ristori. Prima è stato detto che erano pochi ristori per i civili. che in Commissione lo abbiamo evidenziato. In realtà noi abbiamo messo ristori anche per chi ha subito danni sismici, cosa che i precedenti Governi non avevano mai fatto. Perché? Le calamità da eventi sismici sono diverse dalle calamità per eventi alluvionali?

Di notevole importanza è anche l'articolo 6, relativo agli interventi di contrasto al dissesto di versante nei territori collinari e montani: fenomeni che interessano, tra le infrastrutture, anche quelle ferroviarie. La novità è stata proprio quella di inserire nei piani speciali le infrastrutture ferroviarie e questo ci consente di operare con maggiore incisività anche in determinate situazioni.

il blocco di tutta la circolazione su rotaie. Con questo provvedimento interveniamo immediatamente anche su queste situazioni critiche. Poi c'è la situazione dei Campi Flegrei

per diminuire i tempi di approvazione. Quindi, va rivolto un plauso al Governo per aver preso in esame il problema dei Campi Flegrei in maniera così rapida.

Tutte queste criticità hanno imposto la necessità di nuovi interventi organizzativi, procedurali e strutturali, al fine di tutelare il più possibile i cittadini di questa zona così popolosa.

nuovamente il Governo e i Ministri, perché finalmente è arrivato il tempo delle assunzioni di responsabilità. Conosciamo l'Italia, la sua conformazione e le sue fragilità idrogeologiche e sismiche, che abbiamo il dovere di prevenire, e non solo perché in passato si sono spesi molti più soldi per fronteggiare le calamità. Come qualcuno ha detto prima, tra il 2013 e il 2019 abbiamo speso 20 miliardi per le calamità e 2 miliardi per le strutture. Ma il nostro primo obiettivo è prevenire per ridurre i costi, ma soprattutto perché, sopra ogni altra cosa, il nostro obiettivo è difendere la vita e la salute delle persone.

Signora Presidente, i progressi compiuti nel corso degli ultimi quarant'anni per la riparazione dei diritti delle vittime della dittatura civico-militare in Argentina rischiano di essere arrestati dalle azioni avviate dal Governo del presidente Milei in quest'ultimo anno. L'azione per il riconoscimento delle vittime dei *desaparecidos* e la lotta delle Madri di Plaza De Mayo rischiano di essere indeboliti dalle politiche di questo Governo. Eppure dagli anni Ottanta si sono compiute tappe importanti per la memoria: il rapporto *Nunca Màs*, voluto per indagare su migliaia di casi di *desaparecidos* avvenuti durante la dittatura militare; il processo alle giunte militari; le indagini e la ricerca di minori nati da donne sequestrate e tolti loro dalla nascita, oltre all'incorporazione nell'attuale ordinamento giuridico di gran parte dei patti internazionali sui diritti umani, tra cui la Convenzione sui diritti umani. Negli anni Novanta, nonostante l'impunità dei colpevoli, si fecero passi avanti nelle leggi riparatorie per le vittime e per la formazione della CoNaDi, la commissione nazionale per il diritto all'identità. Nei primi anni del Ventunesimo secolo si sono compiuti ulteriori progressi, con la riapertura dei processi contro i responsabili delle morti delle torture, il recupero dei luoghi della memoria, la declassificazione degli archivi della repressione e le politiche educative. È forte, fortissima, la preoccupazione per le iniziative adottate in questi ultimi mesi dal Governo, che mettono in discussione le tappe compiute in Argentina per la politica della memoria. Si affaccia una strategia dell'oblio che passa da due iniziative solo all'apparenza distinte: il licenziamento di milioni di lavoratori pubblici, molti dei quali lavorano nei luoghi della memoria e la decisione di sciogliere il CoNaDi e, quindi, di mettere mettere a rischio la Banca nazionale dei dati genetici, caposaldo per la ricerca dei minori sottratti alle madri. I luoghi della memoria senza lavoratori hanno il destino segnato. Rischiano di essere chiusi. sono la testimonianza materiale di quanto accaduto, della riparazione simbolica per le vittime e luoghi di riflessione e formazione di una cittadinanza consapevole del valore dei diritti umani e della democrazia. Il CoNaDi e la Banca dati sono capisaldi per la ricerca della verità. Invece di raddoppiare gli sforzi per trovare i nipoti, restituire loro la propria identità, le politiche governative rischiano di cessare definitivamente questa ricerca, lasciandoli sommersi nelle bugie e negli inganni della dittatura. Da quest'Aula lancio un appello al nostro Governo, al Ministro degli affari esteri, perché avvii un'interlocuzione col Governo argentino per evitare che il negazionismo si faccia strada. Ci uniamo all'appello delle forze di opposizione argentine, dei movimenti, delle associazioni e dei sindacati per chiedere di invertire questa politica, garantire la continuità lavorativa di tutti i dipendenti pubblici, salvaguardando assolutamente i luoghi della memoria. memoria. *Nunca màs:* così terminò l'arringa del coraggioso procuratore Strassera contro la *Juntas,* i capi criminali del terrorismo di Stato argentino. *Nunca màs,* mai più: questa è la strada che dobbiamo tenere ferma contro ogni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

recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali" stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"